Onorevoli colleghi, comunico che la Conferenza dei Capigruppo estata convocata questa sera alle ore 20, mentre domani sera, sempre alle ore 20, si riunira la Giunta per il Regolamento. Pertanto, le sedute pomeridiane di oggi e domani si concluderanno entro tale orario, anziche´ alle ore 20,30, come in precedenza era stato stabilito.

ha autorizzato una societa, la Po Valley, ad eseguire delle perforazioni, in un ambito di tutela paesaggistica sita nel Parco del Curone in provincia di Lecco, per la ricerca di petrolio. Ritengo alquanto singolare la procedura adottata dal Ministero in quanto, nel totale silenzio, gli enti locali, compresa l’amministrazione provinciale, e si sono ritrovati un piatto servito in tavola a giochi ormai fatti, con il rischio che un’area preservata da numerosi vincoli paesaggistici ed ambientali, esclusa da attivita

il Governo per avere una risposta urgente, rapida e precisa, nella speranza che fatti del genere non abbiano a ripetersi senza che gli enti locali e le amministrazioni provinciali competenti